Per favore, c'è troppa confusione.

L'ordine del giorno reca la deliberazione sul parere espresso dalla 1a Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, in ordine alla sussistenza dei presupposti di necessità e di urgenza richiesti dall'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, nonché dei requisiti stabiliti dalla legislazione vigente, per il disegno di legge: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, recante disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria». Nel corso della seduta dell'8 novembre scorso la 1a Commissione ha espresso un parere favorevole sulla sussistenza dei predetti presupposti e requisiti. Successivamente, da parte del prescritto numero di senatori, è stato richiesto, sul parere in questione, il voto dell'Assemblea. Domando all'estensore del parere, senatore Villone, se intende intervenire.

in tutte queste votazioni la Commissione ha confermato l'esistenza dei presupposti di necessità e di urgenza.

strangolare il dibattito o ad impedire la libera espressione della posizione di ciascuna forza politica e dei singoli commissari.

della maggioranza e del Governo. Scelta, questa, ovviamente legittima, dal punto di vista sia politico sia regolamentare, e che dà ragione di qualche tensione di troppo verificatasi nei lavori della Commissione.

propriamente oggetto del parere di costituzionalità) o di merito e opportunità politica. Entrambi tali versanti, com'è ovvio, non devono, invece, entrare nella valutazione dei presupposti di necessità e di urgenza*, ex* articolo 77 della Costituzione. È ben vero, com'è evidente, che, nell'ambito di un decreto - anche molto complesso, com'è quello di cui ci occupiamo oggi

Da questo punto di vista, dunque, non v'è dubbio che il decreto che andiamo oggi ad esaminare, per ribadire la sussistenza dei presupposti, presenti

ne rende evidente la connessione con il complesso delle scelte che l'Esecutivo sta portando avanti e che la maggioranza sostiene in questo Parlamento. In particolare, è chiara - e ci è stata anche indicata dal Governo in Commissione - la connessione con la legge finanziaria attualmente in discussione.

dal fatto calamitoso, dal terremoto, dall'alluvione, dal disastro, da un'oggettiva e fisica

è chiaro che in questo caso sussistono tutti i presupposti di cui si discute. Tale configurazione del decreto-legge, signor Presidente, non è una invenzione di oggi, sono ormai decenni che tale si rappresenta così nell'esperienza costituzionale del nostro Paese. Non è certamente questo Governo che inventa la condizione da me descritta in questo momento, tale è stata l'esperienza dei Governi precedenti, e anche del Governo che ha immediatamente preceduto questo nella scelta che ha ripetutamente fatto di adottare lo strumento del decreto‑legge.

non nella produzione materiale degli effetti dell'atto normativo. Diversamente, dovremmo ritenere che il decreto‑legge può solo disciplinare fattispecie ad effetto istantaneo per cui o l'effetto si produce nell'immediato, oppure il decreto‑legge non si può adottare. Palesemente, tale posizione non può essere sostenuta. Questa è stata una

accettata e mi sento oggi di ribadire a quest'Aula che bene ha fatto la Commissione a ritenere che essa non fosse sufficiente a negare

per la realizzazione di una fattispecie di qui ad un tempo che deve decorrere, non è argomento che possa indurre a ritenere che il decreto non sia necessario ed urgente; né basta affermare che ci sono possibili profili di incostituzionalità e scelte inaccettabili nel merito, perché le sedi appropriate per svolgere queste osservazioni sono, rispettivamente, quella del parere di costituzionalità e il dibattito in Aula e in Commissione per la discussione, l'esame e l'approvazione. Per tutti questi motivi, signor Presidente,

finestra"). Comunico all'Aula che in tribuna è presente una delegazione del Senato di Romania. Tale delegazione è a Roma per studiare l'attività delle Commissioni di questo Senato nel quadro

Ricordo che nella discussione sul parere espresso dalla 1a Commissione permanente

Si è rimasti ad una valutazione interlocutoria della Presidenza che, proprio in ragione della mancanza di una chiara indicazione normativa, ha rimesso la questione alla Giunta per il Regolamento.

al Presidente del Senato, che poi formulerà la sua decisione in attesa di decisioni di organi collegiali, una questione estremamente importante e significativa. Anche se le parole pronunciate dal collega Villone ci esimerebbero da una valutazione sia generale che specifica, credo che l'Aula debba comunque approfondire i temi. Non si tratta di una volontà ostruzionistica. Gli argomenti sono indicati specificamente e in numero estremamente limitato ancorché il provvedimento,

di portare tale materia ad un approfondimento della Giunta per il Regolamento che ci aiuterà a trovare le posizioni giuste. Ciò non toglie la necessità di chiarire come procedere oggi.

Se l'Assemblea accetta formalmente la decisione di votare per parti separate, procederemo mettendo ai voti, una dopo l'altra,

mi riallaccio a quanto lei ha appena affermato in risposta alla domanda che le veniva dal senatore Pastore: lei, sostanzialmente, ha detto che tutta la materia materia «voto per parti separate» verrà affrontata con riguardo alla sua ammissibilità con un voto da parte dell'Assemblea.

e che riguardano diverse parti separate rispetto al decreto, la votazione sia unica, ovvero vi siano tante votazioni quante sono le richieste di votazione per parti separate, salvo evidentemente quelle assorbite. Faccio presente, Presidente, che, come ella ben sa e come sanno il Segretario generale e i funzionari del Senato, i precedenti del 1994 e del 2006 non sono esaustivi sotto questo profilo, perché in quelle occasioni vi fu una sola richiesta

precedente che si è celebrato in Commissione affari costituzionali proprio con riferimento al decreto in esame, quando il presidente Bianco ha ritenuto di mettere ai voti singolarmente

contrario rispetto ad un unica votazione indipendentemente dal numero, più o meno elevato, delle proposte di votazione per parti separate. Signor Presidente, le sarei grato se alla luce di queste modeste considerazioni

ella ritiene che in presenza di più proposte unica debba essere la votazione, ovvero se le votazioni debbano essere tante quante sono le proposte di votazione per parti separate.

Abbiamo già avuto modo, in quest'Aula, di esprimere apprezzamento per la conduzione dei lavori e vorremmo continuare a farlo, sono però turbato dalla risposta che Ella ha dato al presidente Pastore, le spiego perché. Questa mattina, mi ero informato col Presidente del mio Gruppo, che infatti mi ha autorizzato a porre la questione (evidentemente c'è qualche meccanismo di comunicazione che non funziona), quale mi aveva assicurato che in sede di Conferenza dei Capigruppo c'era stata un'intesa per la quale sarebbe stata consentita la votazione per parti separate, anche perché in fondo, su 188 commi, stiamo parlando di una decina di questioni poste (io, ad esempio, ne ho solo una orale da porre).

come ha correttamente ricordato il senatore Palma poc'anzi. La scorsa settimana, lei ha detto al Presidente della Commissione - e a scanso di equivoci, lo dico al relatore Villone, non c'è un fatto personale nei riguardi del Presidente della Commissione da parte della Casa delle Libertà

Adesso veniamo a sapere, ed è una sorpresa anche rispetto a quella che era stata la ricostruzione che il presidente Matteoli mi aveva offerto, dell'intesa, se così si può definire, in Conferenza dei Capigruppo, per la quale, visto che erano limitate, si sarebbero potute votare le singole parti. Perché c'è questo problema, signor Presidente? Vede, lei ha detto che su questa questione non c'è nemmeno un'opinione certa, perché altrimenti non si approfondirebbe alla Giunta per il Regolamento; allora vorrei che lei evitasse di attribuire sulle sue spalle una grave responsabilità, cioè quella di costringerci a fare una specie di balletto per cui ciascuno di noi parla tre minuti per ognuna delle questioni che vuole porre, alla fine non ci si capisce assolutamente nulla (e stiamo parlando di Costituzione, signor Presidente, di rispetto dell'articolo 77 della Costituzione) e poi si dice all'Aula: «Caldo o freddo non fa niente, vota!». Questo è il contrario di quello che prevede la norma costituzionale. Allora, io la vorrei invitare a riflettere su queste questioni: sono troppe le questioni poste? Sono troppe venti o quindici questioni, vogliamo ridurle a dieci? Va bene, ma non ci tolga la possibilità di far esprimere il Senato su una questione, se questa è convincente, senza essere costretti a votare sull'intero decreto-legge; decreto-legge; poniamo il caso che nel dibattito ci sia il convincimento dell'Aula su una ed una sola questione (quella è la *ratio* dell'articolo 78 del Regolamento), noi stiamo qui rischiando, per l'inevitabile logica che si produrrebbe tra maggioranza e minoranza sul voto che decide se si vota, di lasciare appesi in un provvedimento argomenti sui quali ci potrebbe essere condivisione sulla necessità di uno stralcio, perché magari non si è convinti che quella norma passerebbe al vaglio della Corte costituzionale in caso fosse impugnata. Signor Presidente, è una questione importante, questa; io la prego di consentire ai senatori di poter proporre le posso garantire che non c'è nessuna volontà ostruzionistica: se si arriverà a dieci votazioni sarà grasso che cola, però non ci tolga il diritto di poter far pronunciare l'Aula sulla singola questione, perché altrimenti davvero sarebbe difficile poter andare avanti in una logica di correttezza di rapporti. Noi vogliamo essere corretti con lei, vogliamo avere la possibilità di esporre all'Aula il motivo per cui quella norma non è convincente e di avere un voto dell'Aula che ci dà ragione o torto, ma non ci tolga il diritto di avere ragione o torto a seconda della volontà dell'Assemblea.

la richiesta di approfondimento in sede di Giunta per il Regolamento è legata, al di là delle nostre convinzioni individuali, al fatto che questo problema è stato più di una volta posto all'Assemblea correttezza e buonsenso impone al Presidente, almeno a me come Presidente - le cose le vedo così - di andare in Giunta per avere un chiarimento più approfondito e confrontarci. Per il resto, la normativa e i precedenti mi sembrano assolutamente chiari, perché noi riconfermiamo il diritto pieno,

dove si dice che successivamente nella seduta dell'8 novembre, essendo state concentrate in un numero ristretto le richieste di voto per parti separate sui presupposti di necessità e urgenza, il presidente Bianco ha proceduto alla votazione nel merito di quattro di queste proposte, dopo avere constatato in via preliminare e generale che la Commissione non faceva obiezioni. Quindi, è una conferma della mia tesi: se la Commissione non fa obiezioni. Ho sempre detto che il Presidente di una Commissione svolge anche una certa funzione

e nel pieno rispetto dei diritti sostanziali dei senatori. C'è di più: mi sono preso la libertà di dire che questa illustrazione delle proposte si facesse velocemente prima di passare al voto. Per quanto riguarda questa mattina, si è detto che noi avremmo fatto illustrare le singole richieste; non è che abbiamo parlato di altro, anzi è stato detto che questo voto era un voto che apriva alla procedura per le decisioni di merito. Presidente, mi rivolgo al buon senso suo e dei colleghi del Senato. Che senso ha dare la parola ad un senatore che chiede di votare per parti separate se poi non si mette l'Assemblea

Perché lei ha deciso di dare la parola al senatore che chiedeva la votazione per parti separate, seppure per due o tre minuti soltanto? Per orientare l'Assemblea e per spiegare perché vuole la votazione per parti separate; in due o tre minuti lo fa, dopodiché l'Assemblea si deve esprimere. Diversamente, tanto vale non farlo nemmeno nemmeno parlare, si fa la votazione precedente, ma non è questa la strada che abbiamo percorso, non è questo l'impegno che lei aveva preso. Poi, qui sta accadendo di tutto: leggiamo un decreto dove ci sono norme ordinamentali

ma non stravolgiamo, la prego, signor Presidente, il buon senso perché qui si tratta veramente di buon senso. Poi la Giunta per il Regolamento si riunirà, prenderà tutte le decisioni che vuole, ma allo stato la prego

che quando il provvedimento lo consente ciascun senatore può presentare una richiesta di votazione per parti separate. Su questa richiesta l'Aula o la Commissione votano e se votano... Sì, ma siccome il presidente Bianco, caro senatore Boccia, ritiene che la norma sia applicabile anche in Commissione, mi sono permesso per questo di parlare di Aula e di Commissione. Comunque sia, l'Aula, o la Commissione in via estensiva, vota sulla proposta e successivamente vota per parti separate. Quello che è avvenuto in Commissione, signor Presidente, è semplicemente questo: a fronte di quattro proposte di votazioni per parti separate (in base alle quali si diceva, ad esempio, in una di votare il provvedimento e per parti separate il comma 115, in un'altra il comma 116 e così via dicendo), il presidente Bianco ha posto in votazione l'ammissibilità delle quattro proposte per verificare se la Commissione era o no disponibile a procedere, successivamente, alla votazione per parti separate.

di votare su tutte le singole proposte di votazioni per parti separate; essendo state bocciate le quattro proposte con quattro votazioni diverse, si è poi giunti alla votazione del provvedimento. Quindi, Presidente, non capisco davvero, alla luce di questo importante precedente, la ragione per la quale ella ritiene di dover procedere ad una sola votazione. Infine, lei lei giustamente pone il problema di una possibilità di uso ostruzionistico di questo strumento. Tenga presente, però, che, se lo vediamo sotto il profilo della celerità dei tempi, a fronte di un ridotto numero di proposte per richieste di votazione separata, può verificarsi l'inconveniente di procedere a molte votazioni nel merito ed in ragione dell'accettazione in blocco della proposta di votazione per parti separate, quando magari l'Assemblea sarebbe disponibile alla votazione di una sola proposta. In secondo luogo, Presidente, non ritiene lei che, a fronte della diversità delle proposte di votazione per parti separate, l'Assemblea potrebbe essere indotta a tenere un atteggiamento di mera strumentalità politica e di non soffermare la sua attenzione sulla specificità delle singole proposte? Né può valere il precedente da lei richiamato con riferimento alla proposta fatta dal senatore Saporito perché quella era una proposta unica, con cui si chiedeva di votare separatamente i 25 articoli di un provvedimento.

procedura dell'articolo 102, rispetto dei diritti del senatore, e l'articolo 78, che debbono essere esercitati in maniera corretta. Altrimenti, veramente si scivola verso la possibilità di usare la prima facoltà in cento maniere! Questa è la mia preoccupazione nell'interesse del Senato, non di una parte: non mi innamoro mai di una posizione preconcetta. Ma vi assicuro che gli approfondimenti effettuati vanno in questa direzione.

penso che gli interventi dei colleghi Nitto Palma e Storace, ma soprattutto le precisazioni del presidente Matteoli non siano strumentali,

la condividiamo anche nelle parti in cui, con molta onestà intellettuale, il Presidente ha aggiunto: sia chiaro che questa materia sarà sottoposta all'attenzione della Giunta per il Regolamento. Quindi, la Presidenza sa di aver trovato una soluzione di buonsenso, che deve misurarsi con un ragionamento di attinenza regolamentare. In tal senso, Presidente, condividiamo pienamente sia la sua decisione, sia la sua onestà intellettuale di rimettere la decisione ad una valutazione della Giunta per il Regolamento. Signor Presidente, c'è un elemento di confusione in questa discussione e riguarda tutto ciò che è accaduto in 1a Commissione e tutto ciò che è accaduto in Aula. Se non si fa una netta distinzione tra le procedure di Commissione e le procedure di Aula, tra ciò che il Regolamento prevede per la Commissione e ciò che lo stesso prevede per l'Aula, è inevitabile che si creino equivoci e dissensi. Signor Presidente, in sede referente da sempre le Commissioni organizzano in modo semplificato e sommario - dice il Regolamento - la loro attività. Mi deve consentire di dare un giudizio che ritengo oggettivo: il presidente Bianco ha disciplinato in modo impeccabile e perfetto l'andamento dei lavori della 1a Commissione, sottoponendo perfino alla stessa, e poteva non farlo,

ed è giusto che il Presidente applichi il quarto comma dell'articolo 78, cioè che sia l'Assemblea a decidere se vuole o non vuole che si voti per parti separate. Quindi, tale decisione è impeccabile anche dal punto di vista regolamentare.

assistiamo a una situazione in cui sembra quasi che nella sua decisione equanime sia stata l'opposizione ad aver visto non non accolte le sue aspettative. Signor, Presidente, lei, con molta onestà intellettuale, ha detto che la Presidenza si è presa la libertà di consentire

anche in un contesto di approfondimento della Giunta per il Regolamento, ma restiamo della nostra opinione che l'unica forzatura sia quella di far illustrare questioni che non dovrebbero essere illustrate. Per favore, tutti sono pregati di stare all'essenziale in questo dibattito sull'ordine dei lavori.

anche per un evidente principio di logicità. Non voglio soffermarmi troppo su questioni tecniche, ancorché la semplice lettura del comma 5 dell'articolo 93 del la modalità di votazione sulla questione pregiudiziale, che si effettua in ogni caso con un'unica votazione. Tuttavia, vi è una questione di merito.

la cui urgenza e costituzionalità è stata ben definita dal relatore Villone, che è parte integrante della manovra finanziaria e che ha una sua univocità. Peraltro, non è la prima volta; anzi, più volte il Parlamento ha votato decreti a copertura della finanziaria, anche proposti dopo la presentazione della stessa legge finanziaria. allora, che la richiesta dell'opposizione è palesemente illogica e contraddittoria. Un decreto o è urgente e costituzionale in tutto o non lo è.

Si vorrebbe votare in tal modo sul contratto degli atleti professionisti, sul problema dei veicoli, sul problema delle dogane e delle dichiarazioni telematiche. È evidente a tutti che qui si vuole sancire un principio sbagliato: il voto per

quello che lei ha testualmente detto, riportando il resoconto dei lavori della Commissione. Di fronte alla richiesta, avanzata da alcuni colleghi,

secondo quel prudente comportamento che il Presidente di Commissione non può non avere quando si registra e si cerca di registrare un consenso su una materia così delicata.

Non voglio apparirle insistente...

si renderà conto che si sta introducendo un precedente pericoloso. Sa perché e perché mi sono richiamato all'articolo 129? Lei ha sostenuto, esattamente come il relatore (è un'opinione che rispetto, ma è contraria alla realtà), che siccome un decreto-legge ha un suo percorso unitario, la maggioranza dell'Assemblea deve decidere se si può emendare o meno. Questo significa Questo significa che ha ragione qualunque Governo che, per impedire gli emendamenti, pone la fiducia: ma lo fa il Governo con un atto politico, non è l'Assemblea che proibisce di poter presentare, discutere e votare emendamenti! Qui non ci può essere la fiducia e ci sarà un motivo, presidente Marini, se sui presupposti di costituzionalità non si può porre la fiducia. Ecco perché la invito a riflettere: un solo emendamento, un solo comma vorrei portare all'attenzione dall'Assemblea, e invece nemmeno quello posso fare perché lei, con la sua decisone, ci costringe a chiedere all'Assemblea il voto su tutto, anche se ci fosse una sola norma presuntamente incostituzionale. Stiamo giocando con la Costituzione, lo vorrei dire al presidente Ciampi, al presidente Scalfaro, ai senatori a vita. Con questa decisione

Il punto è un altro ed è stato toccato anche nel dibattito: l'articolo 78 non esclude esplicitamente quello che sto proponendo.

questo io confermo quello che ho detto e poiché il senatore Pastore mi aveva chiesto di esplicitare come dovessimo procedere, ribadisco ciò che ho tentato di spiegare più di una volta:

Signor Presidente, signori rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, io complessiva, in attesa che si definisca la questione della votazione separata che è stata posta, facendo alcune valutazioni di carattere politico e tecnico-giuridico. L'abuso e l'uso della decretazione d'urgenza è un fenomeno che ha ripreso vigore dopo qualche anno dalla sentenza della Corte costituzionale, che ne aveva sanzionato il ricorso improprio. Ne ha fatto uso il centro-destra con recriminazioni del centro-sinistra, ne fa uso oggi il centro-sinistra con la censura del centro-destra. L'articolo 77 della Costituzione da la facoltà al Governo di ricorrere alla legificazione attraverso il decreto‑legge solo in casi straordinari di necessità e di urgenza. La legge n. 400 del 1988 stabilisce i princìpi fondamentali ai quali deve corrispondere il contenuto dei decreti legge, fra cui quello della omogeneità del contenuto Questo decreto-legge viola tutte e due questi richiami normativi. Non c'è la necessità e l'urgenza di tutte le norme, perché alcune entrano in vigore addirittura dopo la finanziaria. Non c'è il contenuto omogeneo perché molte norme del decreto sono disomogenee e incoerenti e alcune hanno una completa estraneità sia al contenuto proprio del decreto sia alla materia tributaria e finanziaria in titolo. Si è detto che il decreto è parte integrante della manovra finanziaria, ma è diventato collegato in seconda lettura e contiene norme estranee a misure a carattere tributario e di riorganizzazione della pubblica amministrazione, al fine di creare quella fonte di copertura di entrata per la finanziaria. Ci sono norme già cancellate dalla micropulitura operata dal Presidente della Camera perché estranee al contenuto proprio, ma altre norme, come: il compenso agli editori da parte di soggetti che riproducono articoli di riviste e di giornali, che entreranno in vigore dopo la finanziaria; il finanziamento per l'acquisto del terreno del teatro Petruzzelli di Bari, che può avere anche precedenti in altri decreti‑legge del Governo Berlusconi,

che la revoca dell'incarico non può essere applicata al personale che viene scelto in base al merito, ancorché a tempo determinato, se non con adeguate motivazioni. Probabilmente sono stati assunti con metodi criticabili, ma con motivazione obbligatoria, come prevede la legge n. 241 del 1990. Pertanto, non possono essere revocati gli atti di assunzione per il mero scorrimento del tempo, cioè dei sessanta giorni previsti. Si tratta di una violazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione, che meglio saranno fatti valere in separata discussione, perché si violano l'eguaglianza dei cittadini in base alla loro collocazione politica e il buon andamento dell'amministrazione. Sicuramente si viola l'articolo 77 perché mancano la necessità e l'urgenza, se non quella di sostituire dirigenti assunti con il centro-destra

La pregiudiziale che l'UDC sostiene, pertanto, ha carattere giuridico-costituzionale e non contenuto prettamente politico che, per quanto di pertinenza, va pure sottolineato. Quindi, si tratta non di rilievi di merito, ma di legittimità. Queste evidenze di carattere costituzionale sono doverose soprattutto perché il voto a favore viene sollecitato a quei senatori a vita di diritto, che della Costituzione sono stati tutori e non riteniamo che lo siano stati a caso o *pro tempore*. Un'altra questione è stata sollevata da un autorevole costituzionalista qualche settimana fa: la violazione dell'articolo 72 della Costituzione, che recita: «Ogni disegno di legge, presentato ad una Camera è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una Commissione e poi dalla Camera stessa che lo approva articolo per articolo e con votazione finale». Tale norma costituzionale è inderogabile per l'approvazione di bilanci e consuntivi. Questo è un provvedimento «collegato», ma certamente si riverbera sull'approvazione di un provvedimento che di articoli ne ha solo due con 181 commi, di cui solo 19 nell'articolo 1 e il resto nell'articolo 2. È evidente che il rilievo costituzionale è sull'articolo 72 e non sull'articolo 77 della Costituzione, ma anche la necessità e l'urgenza devono essere fatte valere con strumenti rispettosi della Costituzione; quella Costituzione che solo alcuni mesi fa è stata difesa dal centro-sinistra nelle piazze d'Italia in occasione del *referendum* sulla riforma della II Parte, attraverso i circoli per la difesa della Costituzione, voluti dal presidente Scalfaro. Non vorrei che, tra qualche anno, dovessimo essere noi dell'UDC a costruire altri circoli per la difesa della Costituzione e della democrazia,

la necessità, appunto, di un voto favorevole circa i requisiti di necessità e d'urgenza, come prevede il nostro dettato costituzionale.

produce una copertura rilevante per la stessa. Inoltre, Presidente, voglio ricordare - come, del resto, ha fatto in modo circostanziato il senatore Villone Villone - che, insieme ai requisiti di necessità e urgenza, dobbiamo prendere in considerazione il decreto al nostro esame

produce quegli effetti che giustificano un voto favorevole circa i requisiti di necessità e urgenza. Da questo punto di vista, mi pare che le norme che dovranno poi essere analizzate ed esaminate nel dettaglio

dal dibattito che si è svolto nell'ultima ora in quest'Aula. Vista la consuetudine che abbiamo appreso dalla finanziaria del 2002, cioè dai lavori parlamentari svoltisi nel novembre e dicembre 2001,

dovesse essere riconosciuto dall'odierna opposizione, che pure ha avuto il merito, perché l'elettorato glielo ha concesso, di governare questo Paese per cinque anni,

Ciccanti, di cui stimo molto gli interventi estremamente competenti in Commissione Bilancio, forse può darmene atto. Signor Presidente, il problema non è scoprire l'acqua calda, cioè scoprire che, quando la vecchia maggioranza diventa opposizione, nega tutto ciò che aveva fatto come maggioranza nel momento in cui le modalità utilizzate dall'odierna nuova maggioranza diventano, guarda caso, le stesse utilizzate in forma di *technicality* dall'allora maggioranza, oggi opposizione.

un Governo emanare un decreto‑legge collegato al disegno di legge finanziaria, del quale l'odierna opposizione oggi registra la mancanza dei presupposti fondamentali di necessità e urgenza? Quale sarebbe il motivo in base al quale i colleghi dell'opposizione oggi registrano l'assenza di quei requisiti? Signor Presidente, io non li ho sentiti; i miei colleghi non li hanno sentiti. I miei colleghi hanno percepito quello che il Paese sta percependo, cioè che la richiesta di un voto sulle pregiudiziali,

organizzativa di lavoro del Governo, che è la stessa utilizzata dall'allora maggioranza, oggi opposizione. non riesco a rinunciare a questo stupore, sarò un neofita della politica e quindi chiedo perdono a tutti gli esperti presenti in quest'Aula, molto più saggi e autorevoli di me. Non riesco a capire come sia possibile difendere un messaggio politico rivolto al Paese, in cui si afferma che questa è una finanziaria durissima, che colpisce soltanto i lavoratori, che nega il giusto diritto alle liberalizzazioni, quello non dovrebbe dire e così via, mentre poi si contesta nel metodo, non nel merito, la modalità che il Governo ha deciso di utilizzare.

di questo decreto-legge. Voglio ricordare agli esponenti più attenti dell'opposizione che all'interno delle Commissioni riunite si è svolto un ottimo lavoro. Lo si sta svolgendo ancora ed è da apprezzare il comportamento di tutti i commissari in quella sede. Noto, in particolar modo, dopo aver letto in questo fine settimana il corposo elenco di ordini del giorno presentato da tutti i componenti della maggioranza e dell'opposizione delle Commissioni riunite, che vi sono notevoli punti di incontro. Voglio segnalare, ad esempio, l'ordine del giorno

condivisibile. È questo modo di pensare che produce la nuova politica: niente da discutere e nulla da recriminare nei confronti del vecchio, ma la disponibilità, l'apertura mentale, l'onestà intellettuale di aprire la mente di fronte alle possibili convergenze, indipendentemente dalla bandiera, dal colore, dal nome del Gruppo

di fronte a situazioni in cui le richieste dell'opposizione odierna hanno coinciso con quelle della maggioranza e viceversa. Oggi, signor Presidente, siamo di fronte ad una situazione in sulla più importante legge del Paese, sulla più importante materia che il Parlamento si trova ad affrontare, c'è la possibilità di guardare con luce nuova questa prospettiva.

quale vi è una brevissima illustrazione delle motivazioni addotte e voglio far presente all'Assemblea che si parla sì, di temi apparentemente minori, ma anche di grandi questioni: lo *spoils system*, l'imposta di successione,

del senatore Ciccanti, per un motivo: noi contrapponiamo la tesi della legalità e della legittimità della decretazione d'urgenza, esposta e suffragata da questo testo, alla tesi della mera opportunità politica o a quella dell'opportunismo politico sostenuto dal relatore, senatore Villone. Egli ha affermato che quello che fa il Governo è sempre ben fatto, che non bisogna cercare le singole norme, ma guardare ad una azione complessiva del Governo. Possiamo anche cancellare la Costituzione ed anche eliminare dal Regolamento del Senato il voto sui presupposti di necessità e di urgenza. Detto questo, signor Presidente, restituisco il microfono.

perché, in tal caso, come ho già detto questa mattina, si innesca quel meccanismo perverso dello scambio o delle vendite delle supplenze, delle ripetizioni private:

Si maschera una serietà facendo cose non serie; allora o si ha il coraggio di farle fino in fondo o si abbia il coraggio di non farle. Questo è il primo punto. Il secondo punto che ci distingue riguarda la terza prova, come ho detto precedentemente. Noi chiediamo che sia una prova che verifichi le competenze dell'alunno e non un esame nozionistico come si vuol continuare a fare, perché l'Europa chiede ai nostri studenti quali sono le loro specifiche competenze alla fine di un corso di studi. Qui si elude ancora il problema, si fa finta di niente; si vuole, con questo piccolo cappello, vestire un manichino che è nudo, perché non esiste una proposta in merito alla alla riforma della scuola superiore. Chiedo al Governo e a questa maggioranza: avete o no una proposta per la scuola superiore? Se l'avete, ditela ditela al Paese e, soprattutto, ditela ai nostri studenti e alle loro famiglie. Si ferma per un attimo la riforma Moratti: posso comprendervi. Ma non si ha il coraggio di dire: non vogliamo quella riforma, vogliamo quest'altra.

serve esclusivamente a dire che abbiamo fatto qualcosa, ma onestamente in questo modo facciamo solo un danno. E non è affatto vero, senatrice Soliani, relatrice del provvedimento, che oggi gli studenti, visto questo disegno di legge (e non so se ne hanno visti altri) stanno studiando più di prima: sono battute politiche, battute di una parte. Vi capisco, vi comprendo, ma sono sciocchezze*. Oggi gli studenti non sanno nemmeno di cosa stiamo dibattendo: questa è la verità, altro che sostenere che sono già più coscienti, che sono sui banchi, più pronti a studiare. Ma stiamo scherzando? Oppure dimentichiamo che la nostra scuola è quella di cui leggiamo in questi giorni sui giornali,

Questo è il problema del Paese: è tutt'altro. Si vuole dare un senso di serietà modificando questo cappello, l'esame di Stato? Per favore, non scherziamo, perché stiamo veramente scherzando. La terza prova rimane quindi nozionistica, antiquata, vecchia, com'è tutto l'impianto che si vuole portare avanti, tant'é che si ripristina un vecchio meccanismo, allontanato da questo Stato da oltre dieci anni.

vedremo se il Capo dello Stato firmerà o meno un disegno di legge così fatto che è chiaramente incostituzionale. La parità scolastica è nella Costituzione; questo Parlamento con la vostra maggioranza ha approvato un disegno di legge sulla parità; se le se le scuole paritarie e le scuole statali fanno parte del servizio pubblico nazionale hanno gli stessi diritti e gli stessi doveri, non sono cose diverse. Gli insegnanti abilitati nell'una sono insegnanti abilitati nell'altra;

Questi sono i tre punti che ci distinguono, e in maniera significativa. Non aggiungo altro, se non una questione ribadisco nuovamente: se veramente avete a cuore la scuola, non si va avanti a piccoli passi.

fatta di conoscenze per i nostri giovani, il Paese non potrà crescere. Non crescerà con questo esame di Stato, perché si vuole far credere agli italiani che, modificando la parte finale di un corso di studi che è quello che è, che tutti quanti conosciamo,

rimettiamo ordine, fate una riforma, se ne avete la volontà politica e se riuscite a trovare un accordo tra di voi, perché sulle scuole paritarie, tanto per dirne una, c'è un disaccordo completo. Sono stati ritirati molti emendamenti, l'ho visto, probabilmente bisogna portare avanti ancora questa maggioranza;

per dare un qualcosa all'opposizione, come qualcuno potrebbe pensare, ma solo perché il disegno di legge governativo forse era stato scritto in maniera molto affrettata e quindi abbiamo sopperito

L'emendamento 1.300 è in sintonia con quel ragionamento di serietà che sia la relatrice, sia il Governo, sia i membri della maggioranza auspicano,

Presidente, l'emendamento 1.30 è stato presentato da Alleanza Nazionale per rendere più seria la valutazione dei cosiddetti ottisti, cioè di coloro che si presentano all'esame di maturità senza avere frequentato l'ultimo anno delle scuole superiori. durante la discussione in Commissione sono stati approvati due emendamenti, uno di Alleanza Nazionale e uno di Forza Italia, che già rendono più severa la disciplina di questo particolare caso e che consentono di migliorare significativamente il testo del Governo. Tuttavia, credo che un po' più di coraggio si poteva dimostrare da parte del Governo, prevedendo una media sicuramente superiore per quanto riguarda le classi precedenti terza e quarta, per andare in quella direzione di maggiore serietà che il Governo e la relatrice hanno più volte vantato e che tuttavia poi nei fatti non sempre è stata seguita. Pertanto, Alleanza Nazionale ripropone questo emendamento come contributo al miglioramento di un testo che tradisce molte delle aspettative che aveva fatto nascere.

Ci sembra molto opportuna una correzione in senso laico di questo provvedimento rispetto all'esame di maturità. Il punto specifico riguarda la

Noi proponiamo semplicemente la soppressione delle parole «o paritario», in maniera che l'esame di Stato torni, com'è logico nel caso dei privatisti, a poter essere effettuato soltanto nelle scuole di Stato.

private riconosciute come paritarie siano abilitate a certificare il corso di studio dei propri alunni, non si vede a quale titolo debbano farlo nei confronti di studenti esterni, che provengano da studi totalmente privati. tratta di un compito che per evidenti opportunità (non direi nemmeno per ragioni ideologiche, ma piuttosto istituzionali) va riservato, a mio modo di vedere, alla scuola di Stato. Per questa ragione voterò a favore dell'emendamento 1.201 e degli analoghi emendamenti successivi.

personale, il mio voto favorevole a questo emendamento per le ragioni esposte dagli oratori che mi hanno preceduto.

Se vogliamo ricordare la legge di parità e se allora non la approvaste tanto per farla o per aggraziarvi il consenso di qualche parte della cosiddetta

da un articolo unico proposto dall'allora ministro Berlinguer. Al comma 4 riportati i requisiti per poter accedere alla parità scolastica: «*a)* un progetto educativo in armonia con i principi della Costituzione (...); *b)* la disponibilità di locali, arredi e attrezzature didattiche propri del tipo di scuola l'istituzione e il funzionamento degli organi collegiali improntati alla partecipazione democratica; *d)* l'iscrizione alla scuola per tutti gli studenti i cui genitori ne facciano richiesta, purché in possesso di un titolo di studio valido per l'iscrizione alla classe che essi intendono frequentare;» (come per le scuole statali) l'applicazione delle norme vigenti in materia di inserimento di studenti con *handicap* o in condizione di svantaggio; *f)* l'organica costituzione di corsi completi personale docente fornito del titolo di abilitazione; *h)* contratti individuali di lavoro per personale dirigente e insegnante (...)». Questa è la legge di parità.

dell'articolo 1 della legge di parità dice (e vorrei che il Governo lo rileggesse qualche volta): «Il Ministero della pubblica istruzione accerta l'originario possesso e la permanenza dei requisiti per il riconoscimento della parità». Se i requisiti non ci sono, il Governo ha tutto il potere di ritirare la parità scolastica a quegli istituti non statali che non si rendono idonei.

Stato e, se non se ne fa un'altra, i suoi argomenti vanno condivisi. Diverso è il problema che viene posto dall'emendamento e cioè se un esterno alle scuole che hanno la caratteristica della parità rispetto a quelle pubbliche

operare una specie di opzione locale o nazionale scegliendo la scuola che gli sembra più utile al fine di un risultato specifico e personale. Io ritengo che la scuola pubblica in questo offra le caratteristiche generali nelle quali ciascuno si può riconoscere e chi, per motivi vari, non ha potuto frequentare la scuola, presentandosi ad una scuola pubblica ha tutti i diritti che ha un qualunque studente che la abbia scelta. Noi indichiamo questa soluzione non per discriminare tra pubblico e privato, ma per consentire una scelta che corrisponde alla pubblicità dell'effetto che una scelta come questa comporta. Quindi, sono favorevole a questo emendamento.

ma anche una partita politica importante che va oltre questo semplice esame di maturità, che nella sua inutilità e nel suo aumento dei costi non può che essere non condivisibile, almeno da parte nostra. campo subentrano in gioco altri valori, altre impostazioni, altri ragionamenti, forse politiche, che adesso fanno parte della maggioranza, su cui nel tempo si sono giocate partite politiche importantissime, fondamentali, che hanno fatto fare al nostro Paese un salto in avanti dal punto di vista dell'integrazione, del completamento della rete del sistema scolastico italiano, perché con quel passaggio della parità, voluta dall'allora Governo di centro-sinistra, voluta e sottoscritta dall'allora ministro della pubblica istruzione Berlinguer (che certamente non era della Lega, tantomeno del centro-destra),

verso la libertà scolastica, verso la libertà delle famiglie di scegliere, verso la libertà dei giovani di formarsi dove e come vogliono, senza interferenza con le scuole di Stato, senza interferenza

Signor Presidente, qui c'è un accanimento non terapeutico, ma contro i privatisti. Perché dico questo? Innanzitutto andiamo ad analizzare la fattispecie del privatista. Indubbiamente c'è anche il privatista che vuole accorciare l'arrivo al diploma (che è vero), ma c'è anche il privatista che il giorno lavora,

sinistra che si rifà all'Europa, sia attenta a quello studente lavoratore che si va a presentare agli esami di Stato. Credo che su questo dobbiamo convenire. Ebbene, Ebbene, in questo emendamento chiedo di modificare il seguente passaggio. Per essere ammesso all'esame di Stato - parliamo delle scuole di Stato, non delle scuole private scuole private - il candidato deve sostenere davanti alla commissione le prove di ammissione. È giusto: deve dar prova delle conoscenze. Ma l'assurdo qual è? È che se

Presidente, in realtà, questa nuova normativa si ispira a due princìpi: è una scelta di classe (e spiegherò perché) ed è una scelta statalista (e spiegherò perché). che l'area cattolica e non statalista della Margherita sia a favore del provvedimento

la scuola statale, e lo fa soprattutto in un Paese in cui la scuola statale il più delle volte, è - quella sì - un «diplomificio». Basta leggere i dati, soffermandosi su che provengono ogni anno nel mese di luglio riguardo i livelli di promozione nelle scuole italiane, per rendersi conto che, se esiste un «diplomificio» in Italia, quello è la scuola

Le statistiche OCSE delineano, per quanto riguarda la scuola italiana, uno scenario più che allarmante: allarmante: non è competitiva, non professionalizza e non predispone nemmeno all'apprendimento. Tant'è vero che lo stesso governatore Draghi, due giorni fa, ha richiamato l'attenzione del Governo

Tanto più che, ormai, in Europa si affacciano classi dirigenti (e non solo, ma anche aree professionali), soprattutto provenienti dai Paesi dell'Est, che

per quanto riguarda alcune aree, tipo il Bangalore) ormai sono competitivi persino con la California e le aree più avanzate degli Stati Uniti. Esiste, quindi, un «diplomificio»

perché spesso le aree più deboli ricorrono alla scuola paritaria, che non è soltanto la scuola intesa come «diplomificio», perché esistono anche scuole paritarie paritarie all'avanguardia. Basti riferirsi, per esempio, ad alcune presenze, non solo a Napoli, ma anche a Milano e in altre grandi metropoli di questo Paese. Contro Contro quelle scuole ci si accanisce per proteggere lo statalismo che ha portato la scuola italiana ai livelli delle scuole sudamericane e del Terzo mondo, statalismo che ha provocato un disastro e ha fatto arretrare il nostro livello di apprendimento. Per questi motivi, signor Presidente, ritengo che gli emendamenti presentati dal collega Asciutti non siano radicalmente contrari a questo provvedimento. Non bisogna, bisogna, cioè, discutere sul fatto che si possa superare la prova di ammissione anche con un'insufficienza, ma sul fatto che la prova di ammissione è una misura discriminante nei confronti delle migliaia di studenti lavoratori che sono costretti a presentarsi da privatisti, perché non possono frequentare la scuola, mentre i figli dei ricchi,

Signor Presidente, questo emendamento era stata concepito come risposta ad un testo originario del Governo che era assolutamente insoddisfacente. Il ministro Fioroni proprio quest'estate aveva sottolineato, addirittura, che il passaggio contenuto nel disegno di legge governativo era volto a favorire l'inserimento degli studenti extracomunitari in Italia; si prevedeva, infatti, un percorso agevolato per gli studenti extra-UE. Ciò era assolutamente inaccettabile, pertanto Alleanza Nazionale aveva chiesto un radicale ripensamento di questa norma. che gli emendamenti presentati in Commissione, in particolare uno della senatrice Capelli, hanno consentito di chiarire la portata del provvedimento, così da non

Sarebbe naturale, normale ed espressione di buon senso che l'anno scolastico in corso si svolgesse con le regole con cui è iniziato:

continua. Sarebbe devastante se dovessimo immaginare di procedere ad una riforma della scuola superiore e poi modificare, per il prossimo anno, nuovamente questa maturità. maturità. Sarebbe veramente un errore molto grave. D'altro canto, le profonde divisioni della maggioranza non hanno consentito l'accoglimento di quelle proposte che pur da una parte di loro sono senz'altro condivise e che la stessa Vice Ministro, in qualche modo, ha anticipato potrebbero costituire oggetto di una riflessione seria in vista di una riforma della scuola superiore. Proprio questo è il senso di questo emendamento, che Alleanza Nazionale voterà convintamente, perché credo occorra uscire dalla logica dell'incertezza e della provvisorietà e dire un no anticipato ad una riforma che rischia di essere transitoria.

le cose: esiste una progressione, un legittimo affidamento, una realtà che collega la famiglia e la scuola ai professori, che ha una sua struttura

che aveva una struttura diversa e che riguardava soggetti che avevano la legittima aspettativa di conservare quella specifica struttura. Ecco perché voterò

in presenza di una situazione che riguardi la collettività della scuola nel suo complesso.

possa tener presente l'intero ciclo di studi, seppure la valutazione deve essere fatta sulle materie prevalentemente del quinto anno. È un emendamento estremamente mite, che non tocca alcun argomento di natura ideologica, né aspetti di natura economica. Risulta veramente difficile capire quale sia stata la logica da parte del Governo e della relatrice di respingerlo, dal momento che si è detto in continuazione che questa riforma serviva a dare un senso a tutti e cinque gli anni delle scuole superiori. Un senso lo acquista, a maggior ragione, se durante l'esame si sa che l'intero ciclo di studi verrà preso in considerazione.

come ho già precedentemente detto, che una delle prove (dico la terza, ma potrebbe essere la prima o la seconda, non è questo il problema) sia una prova nazionale sia una prova nazionale di verifica, che consenta la certificazione delle competenze acquisite. Qui ancora facciamo finta di non capire: se non andiamo a verificare le competenze acquisite da ogni studente e non le enucleiamo di studi, in un pezzo di carta, questi nostri studenti non hanno nulla, non vengono riconosciuti dall'industria, oggi come oggi non c'è più nemmeno possibilità d'assunzione da parte dello Stato, quindi non prendiamoci in giro, anche per quanto riguarda il valore legale del titolo di studio.

farlo. Possiamo continuare ad essere sordi, ma in questo modo non riusciremo a fare del bene ai nostri futuri lavoratori, che sono oggi i nostri studenti, che non potranno accedere alla pari degli altri studenti dell'Unione Europea negli altri Paesi, perché non hanno un attestato dove sia scritto nero su bianco quali sono le competenze raggiunte. Un passo, in parte, in Commissione si è fatto, ma è un passo minimo, è una piccola cosa: noi chiedevamo che l'INVALSI, che è l'istituto nazionale di valutazione, predisponesse una

fra coloro che hanno una concezione moderna di scuola, una concezione di scuola che presuppone la valutazione, dunque la responsabilità, che crede nell'autonomia ma che ritiene che l'autonomia debba essere necessariamente responsabile. allora che un esame di maturità debba anche saperci dare delle indicazioni sulla formazione che è stata effettuata in quella determinata scuola e faccio specifico riferimento a dei dati che credo siano sconvolgenti, che sono stati resi noti a seguito di una indagine proprio di questo istituto, l'INVALSI, di cui ora stiamo parlando e che fanno parte di una ricerca svolta nel novembre-dicembre 2005. Ebbene, pensate, cari colleghi, che con riferimento agli studenti delle scuole medie delle scuole medie italiane, è risultato che solo uno studente su quattro è riuscito ad indicare come si calcola il perimetro di un triangolo, mentre addirittura due ragazzi su tre ignoravano che forma avesse un triangolo rettangolo. Ancora, un ragazzo su tre ha sbagliato un'addizione con numeri decimali, ma la situazione è ancora più grave con riferimento ai licei, alle scuole superiori in generale: uno studente su quattro non è riuscito a calcolare il 30 per cento di 300; sei studenti su dieci non sono riusciti a calcolare l'aumento percentuale confrontando due bollette della luce. Pensate che soltanto il 23 per cento dei ragazzi ha saputo dare una risposta su un quesito che prevedeva di calcolare i tre quinti di 180. 180. Allora, capite che di fronte ad una situazione di questo tipo c'è da chiedersi quale formazione i nostri giovani ricevono nel loro percorso. Dunque dobbiamo, in qualche modo, aiutare anche le scuole a verificare il risultato degli esiti formativi. Dobbiamo aiutare anche le scuole a valutarsi e a responsabilizzarsi.

questa estate aveva chiesto una sostanziale soppressione dell'istituto INVALSI, perché una parte della sinistra, come una parte del sindacato, è profondamente contraria a qualsiasi valutazione delle scuole. Questa estate addirittura avevamo temuto che questo istituto, che pure era stato creato nella XIII legislatura, l'INVALSI, appunto, dovesse essere ridotto ad una sorta di centro studi.

la soluzione che ci viene proposta è una soluzione che la senatrice Capelli di Rifondazione Comunista ha definito pasticciata, un compromesso per cercare di tenere insieme delle posizioni francamente inconciliabili.

fa sì che l'INVALSI possa offrire alle scuole dei modelli che le scuole medesime, nella loro autonomia, possono tranquillamente rifiutare.

quella parte più avanzata della sinistra (penso, come ho richiamato questa mattina, al senatore Polito che certamente non sarà insensibile ad un'idea di valutazione delle scuole, ma per esempio anche al senatore Fisichella che in passato si era sempre dichiarato in favore di una valutazione delle scuole), scuole), a quella parte moderna della sinistra che ha un'idea della responsabilità collegata all'autonomia, chiedo di votare questi emendamenti per dare un segnale di forte rinnovamento. non ha bisogno di un ritorno al passato; con questa riforma, con una riedizione sostanziale di meccanismi già sperimentati e sostanzialmente falliti con la riforma Berlinguer, e con un accoglimento di una parte soltanto delle riforme introdotte dalla Moratti nel decreto delle superiori, questa scuola rischia in realtà di fare qualche passo indietro anziché avviarsi verso quella direzione di forte modernizzazione e trasparenza che noi, nell'interesse dei nostri giovani, nell'interesse dei nostri studenti, chiediamo con forza.

che se fossero stati presi in considerazione favorevolmente dal Governo e dalla relatrice, avrebbero indotto Alleanza Nazionale a votare favorevolmente questo disegno di legge. Mi sento di rivolgere un ultimo appello al Governo ed alla relatrice per riconsiderare le loro posizioni e per anticipare quello che la stessa vice ministro Bastico in Commissione ha dichiarato: noi non siamo pregiudizialmente contrari, ma discuteremo di questa riforma, di questo passaggio, quando affronteremo il tema della riforma della scuola secondaria superiore. Allora, ribadisco: se si vuole veramente progredire in questa direzione non cambiamo ogni anno la riforma della maturità, cogliamo questa occasione,

Presidente, il mio è un appello. Stiamo parlando di esame di Stato, di esame di maturità, dell'esame che definisce la vita scolastica e professionale dei nostri giovani: evitiamo che sia fatto a *quiz*. Il senso di questo emendamento è che vengano evitati, nell'ambito di quella prova,

di una enunciazione troppo sintetica del colloquio nel testo. Mi sono quindi permesso, d'accordo anche con i miei colleghi, di richiamare l'attenzione sulla necessità di un colloquio che sia teso ad accertare i contenuti specifici di tutte le discipline, oggetto del colloquio, e non soltanto un colloquio superficiale come descritto nel disegno, frutto del lavoro del relatore e di altri.

contenuta nel disegno originale. Credo che questo faccia parte di uno spirito, pure contenuto nella finanziaria, quando si dice che si vogliono eliminare le bocciature per cercare di sostenere il bilancio ed il disegno economico del Governo. questo emendamento necessario e da approvare, non certo per agevolare le bocciature - non è questo il nostro compito - ma per portare ad una selezione maggiore, ad una verifica sulla preparazione del candidato.

1.510 vuole dare un contributo per una riforma realmente seria della maturità. C'è da porsi un domanda molto semplice. L'introduzione dei tre commissari esterni è stata motivata dal Governo come un tentativo per avviarci verso una maturità più seria, caratterizzata da criteri di valutazione più rigorosi e oggettivi.

che prevedeva anch'essa la presenza di tre commissari esterni. Ebbene, se andiamo a guardare le percentuali di promossi troviamo che la riforma Berlinguer aveva determinato qualcosa come il 96,4 per cento di La riforma Moratti del 2001, nella sua prima applicazione nel 2002, aveva determinato una percentuale di promossi del 95,7 per cento, per poi attestarsi su percentuali pari al 96,5. È allora evidente che non c'è alcuna significativa differenza per quanto riguarda gli esiti tra le due riforme. Occorre pertanto chiedersi se a questo punto valga veramente la pena di spendere circa 150 milioni di euro all'anno già in un momento in cui questa finanziaria taglia di 3.200 milioni di euro i finanziamenti alla scuola italiana, per fare una mezza riforma e ritornare a una soluzione che aveva dimostrato in passato di non funzionare. Ciò posto, o si ha il coraggio di far sì che tutti i commissari siano esterni tranne un membro di garanzia o piuttosto si lasciano le cose come stanno da questo specifico punto di vista.

Se i colleghi hanno la bontà di seguirmi per due minuti, non di più, parliamo della nomina del presidente di commissione: di legge si dice che i docenti in servizio possono essere chiamati a presiedere la commissione se hanno un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con almeno dieci anni di servizi di ruolo. Perfetto. Andando al punto *f)* l'assurdo è che possono fare il presidente anche i dirigenti scolastici e i docenti *tout*

Vorrei capire perché la relatrice non mi ha risposto, il Governo non mi ha risposto, mi avete solamente negato la risposta. Io chiedo, se possibile, una spiegazione: perché dieci anni li si chiede a chi è in servizio mentre a chi è andato in pensione non si chiede nemmeno un giorno di ruolo?

vorrei appoggiare l'emendamento del senatore Asciutti da noi condiviso in quanto non si capisce perché possano essere riutilizzati i dirigenti scolastici che sono già in pensione quando sarebbe meglio invece utilizzare il contingente in servizio. Tra l'altro, si darebbe anche un sostegno al precariato della scuola e, come ha detto il senatore Asciutti, non si capisce per quale motivo arcano questo emendamento non possa assolutamente trovare accoglimento da parte di una maggioranza che, spiace dirlo, nonostante la nostra buona volontà, si è chiusa a riccio nei confronti delle posizioni dell'opposizione. Noi volevamo migliorare questo disegno di legge, non ci è stato consentito e questo ci dispiace moltissimo.

È già stato detto in altri interventi; è già stato detto in occasione della pregiudiziale; è già stato detto da altri oratori precedentemente, il sistema della formazione e dell'istruzione nel nostro Paese è complesso e variegato. Ci sono stati dei passaggi epocali negli anni passati con il contributo di forze -

con cui si individuano soggetti non statali, *non profit* e non privati che però non sono lo Stato

della didattica, dei programmi, dell'accettazione dei fini istituzionali e costituzionali del nostro Paese, dal punto di vista del diritto del lavoro degli insegnanti che sono ivi ivi impiegati e che in quelle scuole agiscono, dal punto di vista dell'accoglienza di tutti gli studenti. Queste scuole,

lo stesso diritto della legislazione del lavoro per poter fare le stesse cose degli altri e quindi non vedo come possano essere respinti anche questo ultimo tentativo e questa ultima possibilità

vanno a sventolare le bandierine in campagna elettorale, vanno a chiedere i voti, vanno a dire «Noi siamo i vostri paladini, noi siamo quelli che portiamo

aver rinunciato a quel progetto, aver rinunciato a quella presenza politica, essere stati falsi e ipocriti in campagna elettorale. Bisogna essere chiari. Ci tengo che queste parole siano verbalizzate, siano - le ho dette proprio per questo - agli agli atti della Camera alta di questo nostro Stato. Evidentemente, quelle forze politiche che si rifanno a quei principi e che vanno a fare quel tipo di campagna elettorale sono oggi vittime, sono oggi schiave di quella sinistra massimalista, di quella sinistra estrema, di quella sinistra che condiziona questo Governo non solo su questo provvedimento - che è un provvedimento neppure il più importante *(Applausi dai Gruppi* *FI e* *LNP)* anche se riguarda la nostra gioventù, la grande quantità delle nostre famiglie - ma in tutti quei provvedimenti che sono all'ordine del giorno: provvedimenti di ordine fiscale, di ordine

abbiamo anche sentito che gli spinelli, le dosi, le quantità possono essere aumentati. Quella sinistra massimalista, quella sinistra estrema condiziona quelle forze politiche che fanno quel tipo di campagna elettorale, quel tipo di proposta politica - a questo punto - ipocrita e non hanno il coraggio, la forza di distaccarsi da quella situazione, di marcare una presenza, anche solo con un voto di astensione che sarebbe già un passaggio significativo nel contesto di questo di questo provvedimento e di questa situazione che si è determinata in questo momento. Non cade il Governo per un voto di astensione! Sarebbe, però, un segnale importante, l'ultima occasione di questa

senatore Peterlini, ma di scuole serie. Perché dunque non possono queste serie scuole paritarie far sì che i loro dirigenti scolastici possano fare anche i presidenti di commissione? Del resto, ricordo che sono professori di ruolo per la legge sulla parità:

**Il Senato non approva.**

potranno essere membri della commissione esterna anche i supplenti temporanei senza abilitazione. Questo è il ragionamento che fanno sempre i colleghi che parlano che parlano di serietà. Ebbene, l'emendamento 1.176 tende a rendere serio l'esame di Stato, facendo sì che i commissari siano almeno gli insegnanti di ruolo e non supplenti temporanei *tout court*.

ariana, dei supplenti non abilitati e bocciati alla SSIS, possono, anzi devono, nobilitare la scuola statale con la loro presenza. Se questo non è razzismo, cos'è?

Perché vi deve essere questa disparità? Ma come? Stiamo facendo di tutto: le Commissioni pari opportunità e questa maggioranza, così aperta nel volere democraticamente le condizioni uguali per tutti; questa maggioranza che che reclama uguali diritti per tutti! Non capiamo, sul modello di quanto ha detto il senatore Asciutti, per quale motivo i docenti della scuola superiore che provengono dagli istituti paritari non possono essere anch'essi commissari. Che ci venga spiegato! A meno che si debba dire: «aboliamo la scuola privata». Si abbia il coraggio di dirlo. Si abroghi la scuola privata e i diritti decadranno per tutti. Ma fino a quando essa esiste, colleghi, Presidente,

il quale possiamo ragionevolmente modificare questa legge, esattamente laddove, all'articolo 1, è scritto «I commissari esterni sono nominati tra i docenti di istituti statali». Noi aggiungiamo «di scuole paritarie e legalmente riconosciute». Questo punto, che vorrei presentare in maniera estremamente pacata ma ferma, è stato già oggetto della questione pregiudiziale presentata da alcuni colleghi, ma non diminuisce in alcun modo l'importanza e il significato della scuola pubblica. È allora ragionevole il sospetto che è stato manifestato che la contrarietà è esclusivamente di natura ideologica e lo rivela l'emendamento 1.201 della senatrice Capelli, la quale voleva addirittura che gli esami dei privatisti non fossero consentiti presso le scuole paritarie legalmente riconosciute. Chiedevamo semplicemente che con l'accoglimento di questo emendamento si facesse un piccolo, piccolissimo passo avanti riconoscendo una vera e reale parità tra le scuole pubbliche statali e le scuole paritarie. La risposta del Governo su questo argomento è stata estremamente debole: ci si è detto, semplicemente interpretando la Costituzione, che questo oggi non è possibile. Comprendiamo allora il silenzio della relatrice, sia in Commissioneche in Aula. Non vi è stato alcun pronunciamento su questo argomento, almeno nel merito.

che non toglieva nulla alla scuola pubblica statale, ma che dava un'opportunità in più a quella privata. Avevamo anche sottolineato che con la disponibilità dei docenti delle scuole paritarie avremmo costituito con più facilità le commissioni d'esame ricorrendo in misura inferiore a chiamate lontane dalla sede di esame. Quindi, avremmo risparmiato variate decine di milioni dei quali sembrate preoccuparvi molto in sede di esame della finanziaria. È una grande occasione mancata che noi invece non mancheremo di denunciare fuori di quest'Aula.